la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta.

Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero al ricordo del senatore Francesco Bosi, funzionario pubblico, dirigente di partito, parlamentare di lungo corso, uomo delle istituzioni. Francesco Bosi è stato un prezioso interprete dei valori del cristianesimo sociale e democratico, ideali e principi che hanno ispirato e guidato ogni momento della sua vita e che ha difeso con orgoglio in un periodo di profonde trasformazioni dello scenario partitico, qual è stato quello che ha caratterizzato, nel nostro Paese, la fine del secolo scorso e l'inizio degli anni 2000. Dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana, fu, infatti, tra i principali protagonisti di un in progetto di rigenerazione della dialettica politica nazionale in chiave cattolica; un progetto che egli cercò di attuare sia partecipando attivamente alla costituzione di nuove importanti formazioni politiche sia attraverso il suo convinto e appassionato impegno parlamentare; un'esperienza durata ben quattro legislature, di cui due qui in Senato, dove fu anche Segretario di Presidenza. Come Sottosegretario di Stato per la difesa, dal giugno 2001 al maggio 2006, Francesco Bosi seppe distinguersi per rigore, competenza e profondo rispetto per le istituzioni, in un ruolo che gli scenari internazionali successivi agli attentati dell'11 settembre avevano reso particolarmente complesso e delicato. Fondamentale in quegli anni fu inoltre il suo contributo nella piena attuazione della legge sul servizio civile nazionale e nell'approvazione di importanti provvedimenti di natura legislativa, tra cui il decreto-legge in favore dei nostri concittadini civili e militari rimasti vittime di attentati terroristici all'estero. Forte il suo legame con il territorio, con la Toscana e in particolare con il Comune di Rio Marina, sull'isola d'Elba, di cui è stato sindaco per dieci anni. Con Francesco Bosi perdiamo un amico, un collega di tante battaglie parlamentari, un politico appassionato, capace e generoso; la sua incrollabile fede nei valori del cristianesimo sociale e nei principi della democrazia rappresentano un prezioso insegnamento per tutti noi e per le future generazioni. Nel rinnovare ai familiari del senatore Francesco Bosi il cordoglio mio personale e di tutto il Senato della Repubblica, invito quest'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

un collaboratore prezioso, un amico fraterno, un uomo con cui ho condiviso, nella buona e nella cattiva sorte, un lungo percorso politico. Tuttavia, signora Presidente, dopo le sue parole, che sono state così belle e hanno rappresentato così bene la figura del nostro collega scomparso, desidero solo ringraziarla, non solo personale, ma anche della famiglia, perché credo che rimangano scolpite a ricordo di un uomo buono e giusto. Non intendo aggiungere altro perché sinceramente le parole mie e forse anche degli finirebbero per guastare il bellissimo ritratto che lei ha voluto fare

storia di un uomo che ha dato moltissimo alle istituzioni. È stato un uomo di grandi doti e valori, di una rara umanità, sempre pronto a lavorare per il territorio, anche quando ha rivestito incarichi governativi, consapevole del forte legame che lo univa alle realtà locali della Toscana, in cui ha iniziato la sua carriera politica. Perdiamo un grande interprete dei valori democratico-cristiani, una personalità che viveva la politica con passione e impegno e con uno straordinario legame ai principi democratico-cristiani. Proprio in questi giorni i colleghi che con lui hanno lavorato sul territorio in maniera più stretta lo descrivono come l'uomo della mediazione, come un galantuomo sempre disponibile al dialogo e alla ricerca del compromesso. Ecco, a me sembra doveroso ricordare queste doti indispensabili per un buon politico e per fare una buona politica anche oggi. Alla sua famiglia, ai suoi cari, ma anche al Gruppo UDC, che lui stesso ha contribuito a creare, esprimo, a nome di Italia Viva - P.S.I., le nostre più sincere condoglianze.

alle parole del presidente Casini, che ha ricordato benissimo Francesco Bosi, che consideravo e considero un caro amico, una persona molto seria, con un grande attaccamento al suo territorio, a Firenze, all'isola d'Elba e all'Italia tutta; un uomo che ha fatto della politica la propria vocazione. Concludo il mio brevissimo intervento dicendo che vorrei incontrare in quest'Aula tanti uomini come Francesco. Ci ha insegnato tanto e ci può essere ancora oggi d'esempio e d'aiuto.

Presidente, colleghi, la mia esperienza, appena arrivata alla Camera, è stata quella di avere vicino, come compagno di banco, Francesco Bosi. È stata un'esperienza in cui la complessità degli argomenti che via via si affrontavano richiedeva la capacità di operare, dal mio punto di vista, una profonda mediazione tra quella che era la concretezza del tema del disegno di legge che di volta in volta si approfondiva e quello che per me resta un valore ineliminabile del far politica, che era la dimensione profondamente spirituale e profondamente cattolica in tutto quello che si faceva e si diceva; come tenere insieme temi diversi, cercando una sintesi sempre alta, che rendesse omaggio davvero al primato della politica, ma senza che la politica dimenticasse le sue radici. In questo senso, Francesco Bosi è stato un collega molto discreto, molto efficace, molto profondo; una persona a cui non sfuggivano mai le implicazioni anche più sottili di certe decisioni, capace di trovare quel punto di mediazione che nell'apertura verso gli altri - penso effettivamente alla legge sul servizio civile; penso alla presa in carico di tutti i problemi legati alle Forze armate; penso comunque all'esperienza che come sindaco aveva fatto proprio dei problemi del territorio, quindi della massima prossimità ai problemi della gente - trova sempre una sintesi fortemente equilibrata. Quello che colpiva in lui era una capacità di mediazione alta, che io attribuisco in parte proprio alle sue radici democristiane, e nello stesso tempo un punto forte di trascendenza che lo aiutava a vedere i problemi senza mai lasciarsi irretire dalla piccola difficoltà, dall'ostracismo, dalla conflittualità che a volte rappresentano una trappola per tutti noi quando dobbiamo prendere delle decisioni. Era un uomo grande nella sua semplicità, perché era davvero un collega semplice nel formulare i suoi giudizi, nell'esprimere le sue valutazioni, nel dare i suoi suggerimenti; molto rispettoso della libertà e delle scelte di tutti, ma anche molto coerente con il rispetto che pretendeva per la libertà delle sue scelte. effettivamente un uomo politico di cui vorremmo trovare oggi - nella complessità dei problemi che dobbiamo affrontare giorno per giorno - una sintesi alta, laddove la visione della politica non fa non fa mai velo a una visione più profonda di quelli che sono i problemi umani, di quelli che sono i diritti umani; una visione capace di cogliere e declinare l'espressione «diritti umani» nella pienezza del proprio significato, sapendone davvero valorizzare tutta la ricchezza possibile per dare alla vita di tutti noi una dimensione veramente capace di riconciliarci con una visione politica che non è mai mero interesse personale, che non è mai nemmeno interesse del proprio territorio; una visione piuttosto data dall'esperienza probabilmente fatta

Signora Presidente, onorevoli senatori, intanto desidero ringraziarla, Presidente, per le belle parole con cui ha ricordato il senatore Bosi prima come uomo politico; aggiungo le mie riflessioni a quelle fatte anche dal presidente Casini. Francesco Bosi è stato una grande personalità della politica a livello nazionale e - lei l'ha ricordato prima, Presidente - un uomo molto legato al territorio dove ha svolto l'opera di sindaco, all'isola d'Elba, e anche a Firenze dove ha svolto la funzione di consigliere comunale e anche regionale, città che amava molto e alla quale era molto legato. Le sue battaglie sono state tantissime: è inutile stare a ricordarle a lungo perché perché resteranno per sempre importanti nel mondo del cattolicesimo, per i valori che si sentiva di rappresentare. Vorrei ricordarlo anche dal punto di vista personale perché per noi, per il sottoscritto, per molti altri che hanno fatto parte della destra politica, da sempre, sin da ragazzini, Francesco Bosi è stato sempre - anche vedendo le sue immagini - un uomo sorridente, un gentiluomo, una persona per bene. Anche quando era forte il seme della discriminazione nei confronti della destra politica in Toscana, a Firenze, che non era certamente un territorio facile per noi, Francesco Bosi non ha mai fatto sentire questi sentimenti nei nostri confronti; anzi, ci è sempre stato vicino con la sua presenza e dimostrava già da allora di essere una persona perbene. Negli anni c'è stata poi una collaborazione all'interno del centrodestra, tra l'area l'area della destra e il centro che rappresentava quello schieramento politico. Lo ricordo quindi anche dal punto di vista personale e porto il mio cordoglio alla sua famiglia, in particolare al figlio Lorenzo e a tutti i suoi familiari, perché è una grande perdita per il nostro Paese e specialmente per la Toscana e per Firenze. *(Applausi)*.

cordoglio per la morte del senatore Francesco Bosi alla sua famiglia, ai suoi amici e collaboratori, al suo partito di appartenenza. Tra i fondatori dell'UDC, lascia la sua eredità politica di uomo profondamente cattolico, con saldi principi di cristianità e di autentica fede. Ha dedicato il suo tratto umano e gentile alla sua intensa attività politica, che l'ha visto ricoprire ruoli di deputato e senatore, ma anche ruoli legati al suo territorio, la Toscana: come consigliere regionale e poi, a Firenze, come consigliere comunale e assessore. poi, anche la carica di sindaco a Rio Marina, nella splendida isola d'Elba, che ora sarà probabilmente il luogo scelto per il suo riposo eterno. Scompare così una figura umana di piena generosità verso il prossimo, collaborativa e capace di essere, prima che politico, uomo che fa politica. Questa caratteristica, per quanto possa apparire sottile, ancora oggi fa una grande differenza, ed è per questa caratteristica, che è prestigiosa e rara, che lo vogliamo tutti ricordare.

anticipato in vari modi sia in questa istituzione, sia fuori - della calendarizzazione del disegno di legge contro l'omofobia e la transfobia noto come di disegno di legge Zan. nei giorni scorsi due Chiese titolari di una delle intese previste dall'articolo 8 della Costituzione hanno scritto una lettera formale al Capo del Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri,

relativi a materie che coinvolgono i rapporti della Chiesa Apostolica in Italia» (oppure della chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni) «con lo Stato, verranno promosse, previamente in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso». previamente anche nel caso di disegni di legge. Il Senato non può ignorare questo passaggio: le intese sono previste dalla Costituzione, non possono essere modificate con legge ordinaria perché sono equiparabili a un trattato internazionale; possono certamente essere abolite: si abroga la legge e addirittura si abroga l'articolo 8 della Costituzione, che è un presidio previsto dai Padri costituenti per la tutela della libertà religiosa, ma non possono essere ignorate. So che il Governo si è mosso, ma il disegno di legge è indubitabilmente all'esame del Senato. Il Senato non può ignorare previsioni

che, per la cronaca, all'epoca in cui tali intese furono stipulate, era Romano Prodi che ovviamente firmava non per sé ma per la Repubblica italiana. Questa legge impegna tutti noi, perché il Senato della Repubblica - come dice lo stesso nome - rappresenta la Repubblica italiana. Non possiamo ignorare queste cose.

Senatore Malan, terremo conto delle sue osservazioni che si intrecciano

voti la mia richiesta di calendarizzazione con urgenza della mozione per impedire la trattativa e il contratto tra Cassa depositi e prestiti e Atlantia. L'urgenza è dettata dal fatto che è in corso o sarebbe già stato concluso il contratto che, però, contiene una clausola sospensiva dell'efficacia, connessa alla firma da parte del Ministro delle infrastrutture, della transazione che porrebbe fine al procedimento di decadenza. La mozione è volta proprio a impedire che il Ministro firmi. Nel momento in cui dovesse firmare, la mozione diventerebbe inutile e il Parlamento sarebbe messo davanti al fatto compiuto.

o che, comunque, non venga data una risposta esplicita alla richiesta, eventualmente mettendola agli atti, anche per consentirmi di fare ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni. Le solleciterei una risposta sull'istanza depositata. *(Applausi)*.

Eventualmente le cose andassero diversamente dalla sua richiesta, sottoporremo la stessa richiesta che lei ha fatto in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento

in quanto credo non ci sia alcuna affinità tra la libertà di esercitare e professare una religione con le cose di cui ci accingeremo a parlare tra poco. Mi sembra che una persona definita da tutti come il Messia disse di amare il prossimo nostro come noi stessi e, quindi, non mi sembra che le cose evidenziate abbiano alcuna attinenza con il disegno di legge di cui si parlava prima. noi discuteremo la calendarizzazione ed è chiaro che l'argomento che pone o ha posto il senatore Malan si intreccia inevitabilmente con la discussione sulla calendarizzazione stessa, perché costituisce un aspetto di una discussione molto vasta,

lavori». La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi mercoledì 23 giugno, ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori fino al 13 luglio. Nella settimana corrente saranno discussi il decreto-legge sull'assegno temporaneo e, per la seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale sull'estensione dell'elettorato attivo per il Senato. Per la votazione finale di quest'ultimo provvedimento è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Alle ore 9,30 di domani sarà indetta la chiama per la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di due componenti del consiglio di amministrazione della RAI. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 17. Giovedì 8 luglio, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, dell'università e per le politiche giovanili. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito altresì, sempre a maggioranza, che martedì 13 luglio, alle ore 16,30, avrà inizio la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, sul contrasto della discriminazione e della violenza per sesso, genere o disabilità.

Signora Presidente, mi concentro nello specifico sui punti del calendario della prossima settimana. Come tutti i colleghi sanno - perché non abbiamo fatto mistero del nostro operato

certa. *(Applausi)*. Riconosco a tutti i colleghi Capigruppo e ai colleghi che hanno partecipato alla riunione profonda onestà intellettuale nel rappresentare le proprie motivazioni politiche e nel proporre emendamenti al testo del disegno di legge Zan. Come voi sapete esistono, non solamente all'interno di Forza Italia, sensibilità minoritarie e maggioritarie rispetto a questo testo. Questo è il motivo per il quale noi abbiamo chiesto che il provvedimento non venisse

in un percorso di crescita della legge. Come infatti abbiamo detto e qui ripetiamo, riteniamo importante e fondamentale che questa legge venga esaminata; riteniamo vile, sia non portare la legge in Aula, sia portarla in Aula per farla morire e per sgravarsi della responsabilità di averlo fatto, dando la colpa a qualcun altro.

tuttavia, che non possiamo approvare e fare pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* un manifesto, una bandierina, perché in *Gazzetta Ufficiale* si pubblicano le leggi, non le bandierine.

perché si inseriscono in questo provvedimento dei comportamenti che non si capisce se rappresentano o meno un reato fino a che un giudice non dica se lo sono o meno e questa, colleghi, si chiama norma penale in bianco ed è vietata dalla Costituzione. Io lo dico e lo ripeto: voglio la legge Zan in quest'Aula, la voglio a titolo personale e per il Gruppo parlamentare che rappresento. Non voglio, però, una forzatura del tipo «prendere o lasciare». Non voglio essere costretta ad approvare una norma dismettendo i miei diritti di legislatore solamente perché qualcuno mi impone di farlo, privandomi dei miei diritti di persona che rappresenta non solamente le sue intime e profonde convinzioni, ma anche le intime e profonde convinzioni di chi la pensa diversamente. Altrimenti, colleghi, io non sono una liberale, ma una persona che pensa che la mia libertà e i miei diritti siano migliori di quelli degli altri; non è così che si fanno le leggi. È per questo motivo che noi vi chiediamo con tutta l'umiltà, la disponibilità e - ripeto - l'onestà intellettuale che la presenza in quest'Aula ci impone, di riflettere nuovamente sulla mediazione che il presidente Ostellari ha proposto. Ringrazio il presidente Ostellari per la sua capacità di fare sintesi *(Applausi)*, ha lavorato benissimo perché ha messo insieme quello che apparentemente insieme sarebbe stato con grande difficoltà. Colleghi, in questo momento noi abbiamo un testo su cui ci siamo fermati solamente per colpa di una parola; usciamo dall'irrigidimento di posizioni, usciamo dalle bandierine, buttiamole fuori dalla finestra, pensiamo ai diritti delle persone che diciamo di voler proteggere con questa legge e facciamo una vera mediazione al rialzo e non una forzatura al ribasso portando in Assemblea una norma che non è pronta per essere approvata. Colleghi, non è troppo tardi. Se noi in questo momento voteremo un calendario, come voi ci chiedete di fare, che porterebbe in Aula la legge Zan la prossima settimana, è evidente che tale legge sarà solamente quella che voi ritenete debba essere e che quindi debba rappresentare quella parte di mondo che voi pensate debba essere rappresentata in via privilegiata. E gli altri? E la libertà di parola? E la libertà di espressione e la libertà di pensarla diversamente da come voi pensate debba essere inserita un testo in una norma? Colleghi, sono sinceramente convinta che non sia troppo tardi ed è per questo che propongo che anziché forzare il calendario ad una non rapida, ma forsennata, frenetica e folle corsa del disegno di legge Zan verso l'Assemblea la prossima settimana a testo invariato, noi ci si prenda qualche giorno in più. Il presidente Ostellari ha fatto una verifica sul punto; avevamo detto una settimana in più per consentire alla Commissione giustizia, oberata di provvedimenti, che sta già decidendo in congiunta con la Commissione

se non sono solo parole, se noi dobbiamo veramente difendere un diritto, se dobbiamo difendere i diritti LGBTQ cosa di cui io sono profondamente convinta, di cui noi siamo profondamente convinti, non esiste un unico modo per farlo. La politica è mediazione, confronto e capacità di fare sintesi. Facciamo sintesi. Mancava un centimetro alla metà nei nostri tavoli fino ad un'ora fa, andiamo avanti non irrigidiamoci. Non facciamo, collega Malpezzi, salti in avanti eccessivi perché qui non si tratta di vittorie e sconfitte di qualcuno, si tratta di maturità politica di quest'Aula che deve dimostrare di essere capace di rappresentare tutti e non tutti e non solamente una parte preferita. Questo non è parte di un accordo politico che rientra nell'ambito di operatività del Governo. Questa è attività parlamentare. Lo abbiamo detto una volta e lo ripetiamo: il Governo Conte è finito,

di fare della legge Zan una legge veramente condivisa, una legge che sia per noi una prova di maturità politica. Una legge che ci faccia fare ciò per cui siamo qui: lavorare sulle norme per migliorarle. Noi non siamo degli osservatori non partecipanti, siamo dei legislatori, non limitiamoci ad osservare il passaggio della legge Zan senza metterci mano. Lavoriamo insieme per renderla migliore e per migliorare i diritti di chi ci sta a cuore e rappresenta il vero cuore della norma, cioè i suoi destinatari.

Il primo fa riferimento a un caso piuttosto strano, relativo alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. La relazione è stata fortemente voluta dalla sinistra affinché arrivasse in Assemblea ed è stata calendarizzata; dopodiché, all'improvviso, senza che nessuno dicesse o spiegasse nulla, quella relazione è stata ritirata e non se ne parla più. Siccome noi siamo abituati a pensare male, abbiamo l'impressione che qualcuno non voglia che in quest'Aula si discuta dei contenuti di quella relazione, relativa al caso dei gessi rossi in Toscana, perché contiene alcune accuse accuse molto precise, severe e circostanziate nei confronti dell'amministrazione regionale della Toscana e degli enti preposti al controllo. Se siamo noi a pensare male, gradirei che qualcuno della maggioranza si alzasse in piedi e ci confermasse che questa relazione quanto prima arriverà in Assemblea per un voto. Altrimenti noi continueremo a pensare male con più argomenti di quelli che abbiamo oggi, ma sicuramente non taceremo questo fatto.

ha deciso che il bicameralismo non esiste più; quindi non serviva fare il *referendum*, presidente Renzi, perché il PD, con un atto unilaterale, ha deciso che il Senato non esiste più, non serve che lavori, non serve che discuta, non serve che tenti di migliorare un testo. Non serve che i senatori esercitino il loro diritto-dovere di lavorare, ognuno nel proprio campo, per tentare di correggere e migliorare i testi che arrivano alla loro attenzione. La motivazione è evidente. Oltre ai contenuti, che tutti conosciamo, secondo me c'è un altro motivo, un dato politico grande come una casa, signor Presidente, colleghi: all'interno della maggioranza c'è un pezzo di maggioranza che è più maggioranza degli altri e che vuole dimostrarlo. Vuole dimostrare chi comanda all'interno della maggioranza e del Governo Draghi. I padroni della maggioranza sono i 5 Stelle e il PD e lo dimostrano con questo *Diktat*; sono i padroni della maggioranza e si comportano con atteggiamento padronale, con l'arroganza dei padroni di una volta, quindi impongono con la forza dei numeri e dei muscoli a tutto il Parlamento la loro verità, che non può essere contestata. Questo è quanto accade. Come abbiamo detto cento volte e ripetiamo per la centunesima volta che sia questa - è la violenza omofobica, siamo disponibili ancora una volta a ragionare su come rendere esistono - che già esistono! - più severe e più efficaci, se questo è il tema. Temo tuttavia che il tema non sia affatto questo. Noi non possiamo accettare che venga approvata, su una questione così delicata, una norma liberticida (presidente Alberti Casellati, peso le parole: una norma liberticida), che introduce surrettiziamente (ma neanche tanto surrettiziamente) il reato di opinione; una norma che limita, fino quasi ad annullare, il ruolo della famiglia come luogo luogo privilegiato in cui educare i propri figli; una norma che introduce obbligatoriamente nelle scuole di ogni ordine e grado la Giornata della teoria *gender*, persino nelle scuole elementari, persino ai bambini di sei anni. D'altra parte, signor Presidente, come è classico di ogni regime autoritario, l'indottrinamento inizia sin dalla più tenera età; e qui di indottrinamento stiamo parlando. Andate pure avanti come schiacciasassi. Hanno cercato di farvi ragionare e di fermarvi le associazioni cattoliche (ma non ci sono riuscite), le associazioni laiche, quelle femministe, e poi intellettuali Presidente della Corte costituzionale; persino il prudentissimo Vaticano è intervenuto con una nota che non ha precedenti. Ma per voi non conta nulla; conta soltanto la vostra bandiera ideologica da sbandierare; per voi conta approvare una legge, in maniera inaccettabile, in modo tale che voi, che forse - lo vedremo nei prossimi giorni -, siete maggioranza in quest'Aula ma sicuramente siete in minoranza fuori da qui, possiate imporre al resto del Paese, alla maggioranza del Paese, una legge che introduce il pensiero unico e poter controllare chi la pensa in maniera diversa. Questo è il contenuto del disegno di legge Zan e questo spiega l'urgenza e la vostra ottusità nel non accettare critiche e anche messaggi di compromesso o di accordo provenienti dal resto del Parlamento. La nostra opposizione, signor Presidente, sarà molto dura, perché perché non basterà certo - e lo dico anche ai colleghi del centrodestra - modificare una virgola, un punto e virgola, una righina: la legge va modificata nella sostanza

che esiste un'opposizione che si batterà con tutte le forze che ha per evitare questa prevaricazione ai danni del Parlamento e dei cittadini italiani.

la sua richiesta rispetto al calendario è che questo argomento non si tratti affatto? Qual è la sua proposta?

la Commissione sta lavorando e si è in fase di audizione, ma sono sette mesi che questo disegno di legge non è all'attenzione, purtroppo, ma è "buttato lì" in Commissione.

quando si fanno centosettanta audizioni significa evidentemente che si vuole rallentare il percorso del disegno di legge.

finalmente da questo limbo il disegno di legge, che finalmente si mettesse un punto fermo e questo - Presidente, lei me lo insegna - non può che essere, come accaduto altre volte,

incontri al tavolo. Questo tavolo si è riunito già dalla scorsa settimana per ben tre volte, nonostante siamo ancora qui a discutere della calendarizzazione. Al presidente Ostellari

Calendarizziamolo e il presidente Ostellari, che è anche il relatore, perché da Presidente di Commissione si è nominato relatore, ha la facoltà di depositare

chiedendo, ormai da tempo immemorabile, di poter finalmente dare anche al nostro Paese una legge che allarga i diritti. Non è una legge che li toglie a qualcuno:

poi il presidente Ostellari, relatore, deposita il suo testo e la Commissione ha tutte le competenze per poter lavorare e fare un lavoro proficuo, come abbiamo fatto fino ad oggi.

e quindi si tratta anche di scegliere dove vogliamo posizionare il nostro Paese. Io penso che il nostro Paese in Europa debba essere posizionato insieme con i Paesi che sono più esposti sul fronte dei diritti e dell'allargamento dei diritti. Non lo possiamo posizionare dalla parte di chi, come abbiamo già visto anche recentemente, firma documenti che sono esattamente il contrario, cioè la negazione dei diritti.

Questo mette ordine e può avviare le procedure in Commissione per togliere questo disegno di legge dal limbo in cui per mesi è stato tenuto,

orchestrando una campagna di denigrazione. Qui non è un problema di ideologia; il problema è che ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e noi vogliamo assumerci fino in fondo questa responsabilità, votando il calendario e dicendo chiaramente che c'è una data precisa, che è il 13 luglio. In quella data è previsto l'arrivo del disegno di legge in Aula e a quel punto la Commissione finalmente dovrà fissare i termini per poter procedere. C'è tutto il tempo, se uno vuole, per fare un lavoro serio ed efficace e questo risponde pienamente al nostro dovere di legislatori.

tiene a rivendicare il fatto che, dall'inizio dell'avventura in questo Governo Draghi, sia in Commissione, sia di conseguenza in Aula, non ha mai

proprio per testimoniare che sul tema della lotta alle discriminazioni noi ci siamo. *(Applausi)*. Questo è un segnale che abbiamo voluto dare, disegno di legge non lo avete neanche voluto guardare, perché tendenzialmente la logica dice che si abbinano i disegni di legge, si fa un testo unico, lo si porta alla votazione della Commissione e lo si discute. Questo è il metodo, è una prassi consolidata per chi fa parte di una maggioranza.

Ci sono dei gruppi politici che le presentano. Si arriva a un testo che cerca il più possibile di accontentare tutte le istanze. Un testo che noi abbiamo considerato una buona base di partenza. Oggi, nel corso della riunione, abbiamo chiesto ci dato un segnale, da parte del centrosinistra, della maggioranza giallorossa (chiamatela come volete), della volontà di modificare il testo. La risposta che ci avete dato è stata: non se ne parla! Avete rifiutato una proposta di mediazione, fatta dal presidente Ostellari, che teneva conto di tutte le sensibilità.

dovremmo metterci intorno al tavolo a discutere e ragionare senza fretta. *(Applausi)*. Questa era la politica di una volta!

1, la sua proposta pone, come finalità della legge, quanto segue: «La presente legge ha la finalità, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, di offrire la più ampia tutela contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sul genere - perché sul genere c'è dentro sicuramente l'aspetto della transfobia, della lesbofobia e di tutte le questioni di cui avete spesso parlato - e sull'orientamento sessuale, quali espressioni di diritti inviolabili di ciascun individuo, nonché contro ogni forma di discriminazione finalizzata alla disabilità». Ma se questo è l'obiettivo della legge Zan, perché non vi va bene questo articolo? Spiegate perché non va bene.

possibili intenti di buona fede, che sono quelli ovviamente legati a tutelare queste identità. Il rischio vero è che l'obiettivo... per cortesia, così non riesco a sentire niente. C'è troppo brusio.

se, invece, l'obiettivo è introdurre o legittimare la fluidità sessuale e il genere neutro, che sono logiche di mercato, lì noi non ci stiamo! Sull'ideologia *gender* non ci stiamo! Sono logiche di mercato, perché lo sappiamo tutti che, se c'è il genere neutro, è più facile vendere smalti anche agli uomini! Lo sappiamo tutti che è così. Questa è la verità! verità! Queste logiche lasciamole perdere, così come la tutela della libertà personale, la tutela dell'espressione delle proprie idee, sono garantite dalla Costituzione e così deve essere e rimanere. Non ci devono essere reati d'opinione.

ragionare davvero. Mettiamoci lì, troviamo una soluzione, siamo vicini, come ha detto la collega Bernini, e soprattutto facciamo un servizio dando una legge vera ai cittadini e lasciamo perdere le ideologie, che rischiano di fare male al nostro Paese.

non per una sorta di favore personale, di non usare il termine «forzatura» semplicemente perché non è appropriato. Nel racconto di oggi, infatti, la presidente De Petris ha provato a mettere un po' di ordine per dimostrare come il termine «forzatura» non sia assolutamente appropriato, perché al netto di quando

nel mese di aprile, dopo innumerevoli richieste, in Commissione giustizia, dove io mi trovavo perché sostituivo la collega Cirinnà, che in quel periodo era via per

perché c'era una netta contrapposizione con chi ci diceva che di quel tema non bisognava parlare. Non è che noi ieri o la settimana scorsa ci siamo svegliati nel chiedere la calendarizzazione,

le audizioni già svolte alla Camera venissero date per consolidate, conosciute, quindi depositate nuovamente e lette; non ci è stato concesso neppure quello. Abbiamo quindi chiesto che le 170 audizioni potessero essere contenute in un programma molto compatto, in modo tale da consentire alla Commissione di procedere; non ci è stato consentito neppure quello, tanto che da aprile

come spiegava prima bene la senatrice De Petris, avremmo potuto utilizzare altri strumenti per forzare, ma poiché non li ritenevamo corretti, volendo davvero dare il tempo giusto alla discussione, abbiamo provato a rispettare i tempi. Signor Presidente, ricorderà altresì che insieme al presidente Licheri, alla presidente De Petris e alla presidente Unterberger le abbiamo anche scritto, segnalandole le difficoltà dei lavori in quella Commissione, mettendo in evidenza che, qualora non ci fosse stata un'azione, che io voglio ridefinire ordinata, avremmo chiesto la calendarizzazione del provvedimento e non è mai successo nulla. ecco perché, senatrice Bernini, non è una forzatura, ecco perché, senatore Romeo, non è una forzatura, perché stiamo andando avanti da mesi rispetto a questo. Allora abbiamo detto: bene, calendarizziamo, data certa, in modo tale che la Commissione poi lavorerà. Tra l'altro, abbiamo sentito importanti esponenti della Lega dire che bastano dieci minuti per trovare gli accordi. *(Applausi)*. E allora quella Commissione li potrà trovare gli accordi! Oggi scopriamo in Aula che invece non può essere così e sentiamo però anche altre cose che non sono corrette, perché corretto non è neppure il termine "mediazione". Quella che è stata presentata oggi, dal nostro punto di vista (legittimo o meno), non è una mediazione, perché non si può mediare con una proposta che decide di tener fuori dalle tutele e dalla protezione tutte le persone trans o in transizione. Questa non è una mediazione o, almeno, noi non vogliamo mediare su questo. *(Applausi)*. Siccome il presidente

Quell'impianto è completamente antitetico a quello del disegno di legge Zan, per un semplice motivo: esso scardina addirittura la legge Mancino e interviene su una serie di sovrapposizioni che rendono addirittura poco interpretabile la legge che già non abbiamo inventato niente in questo disegno di legge; i termini sono tutti quelli già presenti nel nostro ordinamento e quelli utilizzati dalla Corte costituzionale nelle sentenze. Non solo: non abbiamo inserito un divieto di espressione o limitato la libertà di opinione, perché quella legge non crea nulla di nuovo, estende solo la legge Mancino. Allora diteci se il problema è la legge Mancino; se non volete la legge Mancino, quello è il tema, ma è un altro argomento.

uscita in un determinato modo e resa pubblica. Le informazioni e le posizioni da parte del Governo mi sembrano molto chiare; qui c'entra il Parlamento, non c'entrano le maggioranze vecchie e le maggioranze nuove. C'entra la volontà di dare a questo Paese una legge che questo Paese non ha: estendere le tutele di persone che oggi, per quelle tutele che non hanno, rischiano la vita.

Come abbiamo detto, il disegno di legge di cui si parla, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati (lo voglio ricordare), è qui in Senato da sette o otto mesi (dipende da come li calcoliamo). noi cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo semplicemente di arrivare a una data certa per la discussione in Aula, che ci sembra una cosa opportuna, cosa opportuna, visto il lungo tempo intercorso nello svolgimento dell'*iter* e nell'analisi del testo in Commissione. Potremmo fare magari un parallelismo con l'Odissea: non si capisce chi è Ulisse, chi sono i proci e chi è Penelope perché mi sembra che qui si cucia e si scucia costantemente e continuamente la tela, senza voler mai arrivare al punto.

loro più di tutti dovrebbero sposare i diritti delle persone. Perché di questo stiamo parlando: dei diritti delle persone. Qualcuno ha parlato delle scuole: non c'entra niente, l'autonomia scolastica

ascoltare; evidentemente sono più interessati alla propaganda perché qui viene detto che si tratta di una contrapposizione ideologica. Voglio capire chi in quest'Aula sta parlando di ideologia. Qui stiamo parlando di diritti e chi non riconosce i diritti delle persone

mi sembra che non si voglia arrivare a questo punto, quindi, non c'è altra soluzione. Se poi, come tutti ci auguriamo, in Commissione la discussione sarà

non capiscano di cosa stiamo parlando, o forse lo capiscono bene e stanno facendo una contrapposizione veramente in quel caso per una mera bandierina. Bisogna smetterla con queste posizioni e avere il coraggio di dire in maniera definitiva che i diritti delle persone sono al di sopra di tutto, i diritti delle persone. Non mi interessa se quella persona è un uomo, una donna, un trans o qualsiasi altra cosa; sono persone, ce lo vogliamo dimenticare? Altrimenti di cosa stiamo parlando. parlando. Semplicemente come Gruppo MoVimento 5 Stelle pensiamo che la calendarizzazione del 13 luglio sia opportuna e ci auguriamo che in Commissione si lavori alacremente, energicamente e in maniera seria per provare a raggiungere un obiettivo.

Presidente, vorrei descrivere un quadro che reputo abbastanza diverso da quello che hanno raccontato i miei colleghi negli ultimi due interventi, e cioè la senatrice Malpezzi e il senatore Cioffi. Infatti, quello che hanno descritto loro è un film vero fino alla giornata di oggi, nel senso che hanno raccontato la riunione dei Presidenti di Gruppo di maggioranza, in cui si discuteva

tutto ciò che riguardava due blocchi contrapposti in questo Parlamento che non volevano discutere di un provvedimento che, secondo noi di Italia Viva, è assolutamente indispensabile, ovvero un provvedimento che tuteli contro le discriminazioni omotransfobiche, era un film vero fino ad oggi. Quando noi proponemmo, nel maggio scorso, un tavolo di discussione per trovare una soluzione che mettesse al riparo questo provvedimento, così importante, da voti segreti e da un affossamento probabile in Aula, allora veramente c'era questo scontro frontale fra due coalizioni che non si parlavano, e quindi l'unica strada possibile era quella che la senatrice Malpezzi e il senatore Cioffi hanno descritto, cioè andare in Aula e calendarizzare perché l'altra parte non vuole discutere. Oggi, Presidente, è successo un fatto che io reputo importante e che va valorizzato:

impedirne la discussione, ci ha sottoposto una proposta che per noi è perfettibile, sulla quale vogliamo dire la nostra.

Il MoVimento 5 Stelle, il Partito Democratico e LeU hanno detto no alle ventiquattro ore per votare il calendario per il 13 di luglio. La data certa veniva mantenuta dalla proposta di Ostellari. Erano state chieste ventiquattro ore per votare il calendario mercoledì anziché martedì. È stato detto di no.

non poteva essere il 13 se volevamo far lavorare la Commissione, ma il 20 o il 21 luglio, quindi si trattava di rinviare di una settimana. Anche a questa proposta il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle hanno detto di no. Quindi, Presidente, il film che viene descritto, che parla di una contrapposizione che è rimasta immutata nel tempo e che porta una coalizione a maggioranza a far arrivare un voto sulla calendarizzazione, è vecchio. Oggi, rispetto a una condizione che è mutata, si è deciso comunque di votare il calendario, spaccando la maggioranza che sostiene il Governo Draghi e mettendo a repentaglio la legge stessa. Io, Presidente, non sono preoccupato del fatto che si possa discutere questo provvedimento. Si deve discutere. Sono preoccupato del fatto che così come è stata impostata la discussione in quest'Aula, la legge proposta dal deputato Zan rischia concretamente di non essere mai approvata, sotto i colpi dell'ostruzionismo e del voto segreto.

non pensando che decidendo di affidare la vita di donne e uomini, di persone che dice di voler tutelare "all'incrociamo le dita", sta impostando sbagliata il nostro ruolo di politici, di chi esercita questo ruolo nelle istituzioni pubbliche. *(Applausi)*. Io invito i colleghi del Partito Democratico a tornare in loro stessi, perché non li riconosco, Presidente. Io in quel partito ho sempre riconosciuto il riformismo; ho riconosciuto il dialogo, la costruzione di percorsi positivi e non l'estremismo, che porterà questo disegno di legge a non essere mai approvato. L'invito che rivolgo innanzitutto ai colleghi del Partito Democratico è quello di sedersi e ragionare in tempi rapidi per approvare questo disegno di legge, perché oggi le discriminazioni omotransfobiche ci sono e coloro che le subiscono non sono tutelati dalla legge dello Stato. Presidente, quella legge serve e, pertanto, non possiamo incrociare le dita e vedere come va; non ce lo possiamo permettere. Abbiamo il dovere di approvare una legge avanzata nell'ambito dei diritti. Presidente, noi voteremo a favore della calendarizzazione perché nessuno possa dire che Italia Viva è contraria alla discussione sul disegno di legge Zan, ma l'invito che facciamo al Partito Democratico e al MoVimento 5 Stelle è di smettere di svolgere un ruolo che non gli è proprio - mi riferisco soprattutto al Partito Democratico - per cominciare a discutere nel merito e approvare una legge che serve a questo Stato.

Signor Presidente, vorrei premettere che il Gruppo per le Autonomie voterà a favore della calendarizzazione. *(Applausi)*. Per il resto la vedo esattamente come il collega Faraone.

Il presidente Ostellari oggi, però, ha presentato una proposta valida sulla quale si può lavorare, dove non c'è più questa distanza

a un testo unificato. Penso che, se vogliamo fare del bene alle persone che vogliamo tutelare, cioè le persone che rischiano di essere colpite da discriminazione, dobbiamo

Al contrario, continuiamo a fare la guerra su cose assurde perché sono formalità: se c'è dentro la discriminazione per il genere, ovviamente anche l'identità di genere è automaticamente protetta da questo articolo.

accettando anche concetti che non sono proprio fino all'ultimo quelli che ci immaginavamo, ma che in fondo hanno le stesse conseguenze. Prima di passare alla votazione, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che negli ultimi interventi

La proposta è stata avanzata dal senatore Crucioli, a cui do la parola affinché brevemente ci illustri i contenuti della mozione. Qui oggi non dobbiamo discutere dei suoi contenuti, ma

richiamo la vostra attenzione su questa mozione che ritengo urgente e vi spiegherò i motivi. Innanzitutto, la mozione è stata presentata per chiedere all'Aula di dare indicazioni al Governo affinché non venga firmata la transazione che porrebbe fine al procedimento amministrativo di decadenza della concessione autostradale in capo ad Aspi. Aspi. Qualora la firma della transazione dovesse essere apposta dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si perfezionerebbero anche gli effetti del contratto di acquisto delle quote Cassa depositi e prestiti è in procinto di acquistare da Atlantia: si tratta delle quote che Atlantia ha nella concessionaria Autostrade per l'Italia. È urgente, perché a leggere la la proposta di acquisto delle quote da parte di Cassa depositi e prestiti già accettata da Atlantia - prevede però la condizione risolutiva connessa alla firma della transazione - si evince che che la firma dovrebbe essere apposta nelle prossime settimane, e comunque entro un termine di scadenza ravvicinato. Quindi, qualora dovesse essere firmata la transazione, verrebbe meno l'utilità della discussione della mozione. Pertanto,

di cui stiamo parlando, ovvero il consenso o meno che il Parlamento, rappresentante del popolo italiano, dovrebbe dare nei confronti di una operazione che regalerebbe 8 miliardi ai soci di una società che non è stata in grado di tenere in piedi il ponte Morandi. Ritengo invece che si debba dire al Governo di proseguire nel procedimento di decadenza della concessione, che riporterebbe in mano pubblica la concessione autostradale senza spendere un euro per una rinazionalizzazione doverosa. Questi sono i motivi per i quali vi chiedo di poter calendarizzare oggi stesso o domani o comunque nei primi giorni possibili, atteso anche che il Senato non sta lavorando a ritmo pieno e, quindi, ci sono spazi per la discussione di un tema così importante.

gli interventi di fine seduta, che non sono previsti dal nostro Regolamento: mentre prima erano eccezionali, ora sono diventati un'abitudine.

Signor Presidente, ritengo doveroso intervenire sui fatti che sono accaduti ieri mattina. Nella primissima mattinata di ieri, i Carabinieri e la DIA, coordinati dalla procura della Repubblica, hanno sgominato diversi *clan* dediti al traffico di cocaina. Questo è accaduto nel Comune di Partinico, purtroppo tormentato nella sua storia più recente. Va quindi il più grande plauso al lavoro fatto dai Carabinieri, dalla DIA e dalla procura che li ha coordinati.

Partinico è fatta anche di tanta gente onesta e di tantissimi lavoratori che ogni mattina alzano le saracinesche delle loro attività e vanno nelle loro aziende agricole che sono la base dell'economia locale. Partinico ha bisogno di un riscatto.

Signor Presidente, cercherò di portare all'interesse di questa Aula quello che già il Presidente del Gruppo ha affermato per quanto riguarda la Commissione di inchiesta sulle

di residui di lavorazione che sono stati inseriti all'interno di una *ex* cava per il ripristino ambientale. Nella relazione si scrive, in maniera molto chiara, in maniera molto chiara, che i parametri che consentivano l'accordo per il ripristino della cava sono stati negli ultimi quindici anni in pratica sempre disattesi.

*container* certificati di armamenti e bombe per l'esercito saudita, che verosimilmente lo utilizzerà nella guerra civile in Yemen. Eppure in Italia c'è una legge che che impedisce anche il transito di armamenti verso teatri di guerra o verso quei Paesi che non rispettano le convenzioni internazionali e i diritti umani.

Alvise era una persona molto schiva e infatti non avrebbe mai apprezzato il mio intervento in quest'Aula per ricordarlo, però secondo me è doveroso perché Alvise ha lasciato tanto in ognuno di noi con la sua pacatezza, la sua intelligenza e il suo essere vicino a tutti. Dobbiamo proprio ricordare il fatto che Alvise fosse sempre disponibile per qualsiasi richiesta fosse pervenuta da qualsiasi cittadino in difficoltà. Ci ha aiutato moltissimo nel risarcire i cittadini colpiti dalla crisi delle quattro banche, per poi proseguire con il Fondo indennizzo risparmiatori; ci ha permesso di trovare 1,5 miliardi per indennizzare tutti questi risparmiatori e abbiamo fatto veramente un lavoro immane con lui. Non aggiungo altro. Era una persona molto intelligente e al contempo molto schiva, come ho detto prima.

Signor Presidente, quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere ha dell'incredibile. Sembra che ci sia un altro mondo, quello carcerario, così vicino e così lontano dai diritti umani. possibile che tali atrocità si consumino in uno spazio eminentemente statale e per mano di uomini dello Stato? Provo sconforto e sconcerto per fatti così gravi, che hanno portato all'emissione di 52 misure cautelari

In diverse circostanze ho sollevato la necessità anche di costituire una Commissione di inchiesta sulla condizione delle carceri, con riscontro purtroppo negativo. Ho visitato le carceri e ho sentito dalla viva voce dei detenuti lo squallore di quanto sono costretti a subire, al di là di ogni ragionevolezza. Aggiungo altresì che, se questo caso è rimbalzato all'attenzione pubblica, è perché le telecamere distrattamente - come riferisce qualcuno - erano state lasciate aperte. Ma un'ulteriore precisazione va fatta: trovo squallido strumentalizzare politicamente il reato di tortura, su cui adesso ci sono solerti mobilitazioni, anche con ipotesi di *referendum* a ridosso del semestre bianco e quasi a due anni dalla fine della legislatura. E chissà perché, mi chiedo, quando le stesse persone, che vivono questo Palazzo da decenni, non hanno fatto alcunché, salvo aggravare la situazione carceraria. Adesso attribuiscono la responsabilità all'ex ministro Bonafede e all'ex sottosegretario Ferraresi. Semmai, è noto il loro tempestivo intervento per accertare i fatti, nel pieno rispetto delle regole e delle loro prerogative. Come cittadina, come parlamentare e senatrice del MoVimento 5 Stelle, manifesto la mia solidarietà ai detenuti vittime di violenza e alle loro famiglie. I diritti dei cittadini non si toccano e non si toccano i diritti dei cittadini detenuti, dei quali lo Stato per primo dovrebbe garantirne il rispetto.